9,31).* Colleghi, ricordo che, in seguito alla ripetuta mancanza del numero legale, la seduta antimeridiana di ieri

Ieri abbiamo tolto dalla Costituzione la pena di morte; oggi ci apprestiamo a trattare una legge sulla tortura. La settimana scorsa abbiamo affrontato il tema della Birmania, che oggi è di estrema attualità. Proprio per questo vorrei richiamare l'attenzione dell'Aula rispetto a quello che sta succedendo oggi a Rangoon. Il peggio, ciò che temevamo, sta accadendo. Le notizie ultime che provengono dalla Birmania ci parlano di una furibonda repressione contro i monaci e i giovani che ormai da tempo scendono in piazza.

con la delegazione italiana che è a New York, per far sì che il Consiglio di Sicurezza possa affrontare il prima possibile il tema. Chiediamo soprattutto che il Governo italiano faccia subito sua un'iniziativa relativa a un embargo a sanzioni commerciali nei confronti del Governo birmano e, da ultimo ma non da meno, che a livello europeo finalmente si prenda una posizione più dura e rigida all'interno della posizione comune.

altresì assolutamente imperativo che il Governo annulli l'invito fatto ad alcuni rappresentanti della giunta militare birmana a partecipare prossimamente a un incontro di formazione sui diritti umani in Italia: ciò, alla luce dei fatti, mi sembra perlomeno paradossale. Ringrazio il Presidente per la disponibilità a riaprire la discussione. Cerchiamo di vedere come sia possibile scambiare ipotesi di lavoro con il Governo, considerati i recenti sviluppi.

nell'esprimere rincrescimento sul fatto che il Governo avesse reso meno incisivo il dispositivo della mozione. Ciò si poteva capire per le esigenze diplomatiche e per le relazioni, che il Governo ha posto come giustificazione a questa modifica della mozione. Tuttavia, i fatti di oggi dimostrano che occorre un'azione immediata di richiamo da parte del nostro Governo verso le autorità birmane e la loro rappresentanza in Italia.

i fatti che avvengono in queste ore nell'ex Birmania richiamano l'attenzione del Parlamento e di quanti credono vivamente nei valori della libertà e della democrazia nei riguardi di una dittatura militare spietata, che ha un rapporto preferenziale con la Cina comunista e con quei rapporti a livello internazionale. Credo che da parte del Governo italiano ci debba essere un'attenzione particolare, anche perché le Nazioni Unite in queste ore stanno richiamando alla responsabilità. C'è l'attenzione di tutto il mondo libero nei riguardi delle manifestazioni e si pensava fino a ieri che, davanti a tale attenzione, la dittatura militare non sarebbe scesa in campo. In queste ore l'arresto di tanti bonzi e di tanti cittadini dell'ex Birmania testimoniano che quella dittatura chiusa in se stessa non ha intenzione di ascoltare

un pericolo molto più vicino a noi. Questa mattina, passando davanti al Ministero della giustizia, in via Arenula, memore anche dei richiami del Governo

La seduta è ripresa;

questi aspetti tecnici dei quali si discute, in modo da essere pronti per una sollecita ripresa dell'esame in Assemblea.

definitiva valorizzazione, deve conoscere un'ulteriore fase di sistemazione per rispondere alle osservazioni presentate dalla 1a Commissione, che rivela alcune contraddizioni con la legislazione vigente, e anche per rendere questo strumento realmente efficace alle diversità esistenti nelle realtà territoriali, dai piccoli ai grandi Comuni, che non si presterebbero ad essere normate da uno strumento rigido.

Presidente per aver chiarito che l'attuale confusione è determinata da richieste dei Gruppi di maggioranza; quindi, il senatore Boccia

Poi, fortunatamente, si è rinsaviti e si è discusso proficuamente sui vari aspetti, accogliendo i pareri delle altre Commissioni interessate.

Si è constatato da tutti i Capigruppo, me compreso, che i provvedimenti all'ordine del giorno dell'Assemblea non avrebbero comportato questioni pregiudiziali particolari e che tutti i problemi sarebbero stati risolti in Aula. Per questa ragione preannuncio il voto contrario dell'UDC a qualunque rinvio in Commissione di qualunque provvedimento all'ordine del giorno, compreso quello sullo sportello unico,

Le motivazioni dei colleghi Allocca e De Petris non sono assolutamente convincenti. Il dibattito in Commissione è stato esauriente e si è arrivati ad un accordo complessivo sul provvedimento, migliorandolo sotto molti aspetti, compresi quelli segnalati dalla collega De Petris. Il fatto che non ci sia il parere della 13a Commissione mi sembra irrilevante. Moltissime volte le Commissioni non rispondono con tempestività alla richiesta di parere della Commissione che sta

Onorevoli senatori, il disegno di legge in esame differisce di diciotto mesi il termine, scaduto il 4 settembre 2006, previsto dall'articolo 4 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per l'esercizio della delega relativa all'istituzione degli Ordini delle professioni sanitarie, infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione. L'atto è stato esaminato in sede referente dalla Commissione igiene e sanità, che lo scorso 25 luglio mi ha conferito, all'unanimità, il mandato a riferire in senso favorevole sul disegno di legge, nel testo licenziato in prima lettura dall'altro ramo del Parlamento. Quanto ai contenuti della delega, giova ricordare che il richiamato articolo 4 della legge n. 43 del 2006 ha conferito una delega al Governo sulla base di determinati princìpi e criteri direttivi, tra i quali in particolare: la trasformazione dei collegi professionali esistenti in ordini professionali, con l'istituzione di un ordine specifico per ciascuna delle citate aree di professioni sanitarie e con un'articolazione in albi separati per ognuna delle professioni previste; la possibilità di costituire un unico ordine per due o più delle aree di professioni sanitarie individuate; l'eventuale istituzione di ordini separati per le professioni i cui albi abbiano almeno 20.000 iscritti; l'aggiornamento delle figure professionali da includere; l'articolazione degli ordini, a livello provinciale, regionale o nazionale, in relazione al numero degli operatori. In considerazione dell'opportunità di consentire al Governo di procedere al riordino del settore nel senso indicato dalla legge n. 43 approvata nella scorsa legislatura, esprimo l'auspicio di una sollecita approvazione definitiva nel medesimo testo licenziato dalla Camera dei deputati.

voterà a favore di questo disegno di legge che riguarda esclusivamente, come ha detto la relatrice Binetti, il differimento dei termini per l'esercizio della delega. Vorrei ricordare a quest'Aula che la legge delega, che riguarda l'istituzione degli Ordini delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, è stato approvato dal Parlamento al termine della XIV legislatura;

nei termini previsti dall'articolo 4 della legge del 1° febbraio 2006, gli appositi decreti legislativi.

questo decreto legislativo che passerà poi per le apposite Commissioni parlamentari; esso, soprattutto, darà una risposta a quelle categorie impegnate nelle professioni sanitarie che da tanto tempo aspettano di avere una soluzione per quanto riguarda la loro definizione professionale. Ecco le ragioni e i motivi per cui è urgente che il Parlamento, in questo caso il Senato, approvi il disegno di legge.

intendo soltanto associarmi alla posizione del senatore Iovene per dire quanta fretta c'è nell'approvazione di questo provvedimento, perché tutte le professioni sanitarie attendono questa risposta da tempo.

Signor Presidente, l'articolo 1, come giustamente ha detto la collega Binetti, definisce l'ambito di applicazione del provvedimento e rinvia, ai fini dell'individuazione delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie al decreto ministeriale del 2001, adottato in attuazione della legge n. 251 del 2000, specificando che le professioni sanitarie sono quelle che svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione. È fatta salva la possibilità, ovviamente, per le Regioni, di individuare

chiediamo che, in sede di esercizio della delega per l'istituzione degli ordini ed albi professionali delle professioni sanitarie, il Governo proceda all'adozione di uno o più decreti legislativi a carattere settoriale e recanti disciplina organica della materia. chiediamo che venga indicata una disciplina organica della materia proprio per evitare - lo dico da federalista convinto - che in qualche modo le Regioni possano riconoscere come ed albi anche professionalità che magari tali non sono. Faccio un esempio: nei nostri ospedali oggi è riconosciuto come infermieristico personale da cui mi auguro di non essere mai curato. Addirittura adesso abbiamo una serie di infermiere provenienti dal Maghreb che per motivi religiosi lavorano con le mani coperte, perché devono coprire anche le mani. Queste persone curano i malati, li accudiscono, vengono a contatto con parti nobili e non nobili;

accade a livello pratico. A livello poi di conoscenza, vorrei sapere chi controlla, per esempio, che il medico che viene dal Guatemala

come Gruppo di Alleanza Nazionale esprimeremo il nostro voto favorevole a questo provvedimento. Tuttavia sarebbe opportuno che l'Aula sapesse fino in fondo la verità, perché poi, alla fine,

Sarebbe opportuno che qualche collega, anche di quest'Assemblea, si rileggesse gli interventi che fece all'epoca, sia in Commissione che in Aula, dicendo che si trattava di un provvedimento urgentissimo. Già oggi immaginare che si vada ad un differimento ulteriore significa prendere ulteriormente in giro queste categorie che si aspettavano ben altro dal Parlamento. Tant'è vero che il ministro Livia Turco, appena insediata, correttamente, sulla base della legge n. 43 del 2006, preparò quattro decreti attuativi della stessa, per la trasformazione di questi collegi

Resta il fatto che queste categorie sono particolarmente sorprese dall'atteggiamento di un Parlamento che nel 2006 all'unanimità, o quasi, ha approvato

ricordando a qualche immemore senatore che è opportuno che si rilegga le cose che ha detto e gli impegni che ha assunto in quella sede, oltre che, pubblicamente, in una serie di assemblee indette con queste categorie professionali,

sul fatto che il bene salute è custodito in modo molto attento, anche sotto il profilo della procedura del riconoscimento dei titoli di studio dei professionisti che vengono dall'estero.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo Insieme con l'Unione-Verdi-Comunisti Italiani voterà

che l'istituzione di nuovi Ordini (in particolare quando riguardano le professioni sanitarie, infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, vale

Credo, peraltro, che vada anche tenuto presente il fatto che in questo momento siamo di fronte ad una delega di riordino complessivo degli Ordini professionali e che quindi non possiamo proseguire con il riordino delle professioni sanitarie in modo slegato da quei princìpi che devono garantire uguaglianza fra tutte le professioni. Penso, in particolare, al fatto che gli Ordini hanno un senso quando rappresentano uno uno strumento di garanzia rafforzata per i cittadini e prevedono opportune articolazioni al loro interno in albi professionali, il che non mi sembra sia previsto per tutte queste professioni sanitarie.

se prevista - per l'appunto - per chi lavora nel settore pubblico, perché i pubblici dipendenti sono già obbligati al rispetto di codici di comportamento che costituiscono parte integrante dei contratti collettivi e dei contratti individuali che ciascun dirigente rinnova periodicamente con la propria amministrazione. Pertanto, come Gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea preannunciamo il voto favorevole su questo provvedimento di proroga, perché pensiamo che il Governo debba avere il tempo sufficiente per esercitare la propria delega. Ricordiamo però che abbiamo grandi perplessità sul merito, e che quando l'esercizio della delega del Governo arriverà nelle Commissioni, in particolare nella 12ª Commissione di merito, riguardo alle professioni sanitarie, saremo molto attenti che non ci sia una proliferazione di ordini. Saremo attenti che tali ordini, come spesso succede, non abbiano

l'adeguamento alla disciplina comunitaria delle professioni sanitarie. Abbiamo avuto una serie di audizioni con i rappresentanti di tutte queste categorie. Anche in quella sede, ho dovuto riascoltare l'ennesima presa di posizione da parte dei Gruppi parlamentari di maggioranza che hanno ribadito: state tranquilli perché tutto sarà a posto. Bastava chiudere gli occhi e si era di fronte allo stesso scenario dello scorso anno.

meritato lo scorso anno, con una legge votata dal Parlamento, un atteggiamento diverso. Ci auguriamo che si proceda in tempi abbastanza veloci a fare in modo che questi collegi diventino ordini professionali e che sia dato riconoscimento a queste categorie che servono la sanità in maniera seria, avendo acquisito professionalità attraverso titoli di studio particolari, da triennali o addirittura a quinquennali in alcuni casi. Soprattutto, essi hanno un ruolo importante all'interno delle strutture sanitarie, e tutti noi

a ben pensare, ci può essere una volontà di perfezionare l'attuazione della delega oppure quella di cambiare la legge, ossia di inserire

meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso ad Ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi una riduzione di quelli già previsti - dalla legislazione vigente, e non si capisce quindi come facciamo a farne dei nuovi favorendo, il ricorso ad associazioni, di cui all'articolo 8, per ordini, albi, e collegi già esistenti, per i quali non ricorrono specifici interessi pubblici che rendono necessario il ricorso al sistema ordinistico. In

l'assoluta necessità di eliminare una fortissima discriminazione, anzi un'ingiustificabile discriminazione, ai danni di quelle professioni che non avevano a disposizione un ordine precostituito, proprio. Stiamo parlando di oltre 150.000 professionisti.

professionisti avevano creduto a questo tipo di lavoro; avevano creduto che qualsiasi Governo avrebbe compiuto quegli adempimenti necessari affinché il loro riconoscimento diventasse effettivo. Ciò anche perché il Parlamento aveva riconosciuto questa assoluta necessità.

il passaggio, non è che la pratica sia rimasta dimenticata nel cassetto del Ministero della salute: c'è stato uno scontro fortissimo, ideologico e culturale, all'interno della vostra maggioranza, all'interno del Consiglio dei ministri, tra il ministro Turco e il ministro Bersani.

professionisti che sono stati dileggiati ben due volte. A questo punto non so se il Governo riuscirà ad onorare questo impegno, ma per noi questa è l'ultima scadenza. Dopodiché siamo anche disposti a fare le barricate, perché questa è una ingiustificabile discriminazione a danno di professionisti che, tra l'altro, svolgono professioni estremamente delicate e che, proprio perché la loro presenza a livello territoriale e professionale è così importante, crediamo debbano essere assolutamente aiutati e valorizzati

varata sì dal Governo di centro-destra, ma che allora vide la partecipazione di tutti, ad eccezione di Rifondazione Comunista, in una votazione all'unanimità.

di volta in volta abbiamo cercato di riconoscere la professionalità raggiunta. Il mondo della sanità è composto, sicuramente da medici, ma anche da tante altre professioni sanitarie, tra le quali quelle di cui stiamo parlando, cioè infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie

cercato di portare avanti all'unanimità. Del resto, tutti i partiti in questi giorni hanno incontrato le delegazioni, garantendo al massimo l'appoggio per questo provvedimento. Invece, oggi, che cosa troviamo? Troviamo una situazione quasi

quando si viene stimolati, quando si viene tirati per i capelli o per la giacchetta, come avete fatto voi, invece di affrontare il discorso in modo sereno e tranquillo. Io sono a conoscenza che, in alcune Regioni, anche questo slittamento, questa scelta dei decreti delegati risentono della lotta per il Partito democratico,

state bloccando la Nazione per una lotta tra partiti! Oggi eravamo d'accordo con voi, eravamo pronti a votare all'unanimità, eppure avete cercato di mettere una foglia di fico per nascondere le vostre vergogne. L'Italia è bloccata dalla vostra lotta di potere! *(Vivi*

Signor Presidente, onorevoli colleghi, spero di riportare un po' di serenità e di calma nella discussione. Il provvedimento che ci apprestiamo a votare reca la proroga fino al 4 marzo 2008 per l'esercizio da parte del Governo della delega prevista dalla legge n. 43 del 2006, per l'istituzione degli Ordini e degli albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione. Credo sia giusto dire che questo provvedimento di proroga non è legato ad una disattenzione del Governo, ma ad un atto di coerenza; la proroga, infatti, si rende necessaria al fine di collegare la regolamentazione delle professioni sanitarie non mediche nell'ambito del più ampio provvedimento di riforma di tutti gli ordini professionali attualmente all'attenzione del Parlamento, affinché tutto il settore abbia un indirizzo omogeneo ed uniforme. Il contenuto della delega consentirà anche alle professioni sanitarie non mediche di poter contare su un'organizzazione capace di soddisfare le necessità di valorizzazione e di tutela delle specifiche professionalità, che nel nostro ordinamento sono state individuate nel numero di 22, nelle varie aree della sanità. Ma soprattutto l'istituzione di ordini o di albi anche per queste professioni, che verrà fatta nel rispetto delle direttive europee sulle liberalizzazioni e sulla libera circolazione dei professionisti, non deve essere vista come un moltiplicarsi di corporazioni, ma piuttosto come un contributo valido, e direi indispensabile, per la garanzia della qualità professionale degli operatori del settore e, soprattutto, come una maggiore tutela e rassicurazione per tutti i cittadini, in un campo così delicato, quale quello della salute umana, nel quale la qualità della prestazione offerta è elemento basilare ed irrinunciabile. Altro punto di grande interesse riveste la formazione professionale: tra i requisiti essenziali previsti per l'esercizio di queste professioni sanitarie, è infatti richiesta un'abilitazione rilasciata dallo Stato, in seguito al superamento di specifici corsi universitari, in linea con la normativa europea in materia di libera circolazione delle professioni, e pone il nostro Paese in posizione di avanguardia nel panorama europeo nell'ambito delle professioni sanitarie. Concludo sottolineando che in questo momento particolare, nel quale stiamo affrontando una revisione dell'intero assetto del Sistema sanitario nazionale, per un suo necessario ammodernamento, l'intenzione - che ribadisco assoluta - di valorizzare le professioni sanitarie, evidenzia il ruolo fondamentale delle stesse nell'organizzazione e nel funzionamento del sistema socio-sanitario del nostro Paese. Tutto questo nell'ottica di quello che deve essere il nostro obiettivo primario: la tutela della salute delle nostre comunità come bene primario, in ossequio al dettato costituzionale. Per questi motivi il Gruppo de L'Ulivo voterà con convinzione a favore del provvedimento, con l'auspicio evidentemente che i tempi della delega possano anche essere abbreviati. *(Applausi

offrire al Paese la convinzione certa che l'intero Senato da un lato fa propria la tutela della salute dei cittadini e dall'altro, per tutelare questa salute, garantisce i professionisti della salute nel rispetto dei loro diritti e nella richiesta di un codice deontologico alto, forte, sicuro ed esigente. Per questo chiederemo che che tale tipo di provvedimento abbia un suo percorso privilegiato adeguato al bene che tutela.

Presidente, vi è stata una richiesta di rinvio in Commissione.

di mezz'ora, in quanto il provvedimento è stato lungamente discusso in Commissione, c'è stato un contributo di tutti i Gruppi politici ed è possibile vi sia qualche punto di ulteriore miglioramento. Vorremmo dunque verificare se in questa mezz'ora sia possibile trovare un'intesa sul modo di procedere.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge oggi al nostro esame nasce dall'esigenza di semplificare, razionalizzandole, le procedure amministrative che intralciano il percorso di un aspirante imprenditore nel momento in cui decide di avviare un'attività d'impresa. Il provvedimento contiene una disciplina finalizzata alla semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese attraverso lo snellimento dei procedimenti di competenza dello Sportello unico per le attività produttive, con riduzione dei relativi termini e una più ampia autorizzazione della autocertificazione e della dichiarazione d'inizio d'attività. Oggi nel nostro Paese chiunque decida di voler avviare un'attività d'impresa si trova imbrigliato in una fitta ed intricata rete di trafile burocratiche, pratiche amministrative ed autorizzazioni. Si tratta di un vero e proprio supplizio, che rischia di imbavagliare e di soffocare lo slancio innovativo dell'imprenditore stesso. Le idee, soprattutto quelle dei giovani imprenditori, rischiano di restare schiacciate dalle strutture burocratiche, con grave danno per la collettività e lo sviluppo economico. Secondo studi effettuati a livello europeo, i tempi necessari per far decollare in Italia un'impresa possono arrivare fino a 35 giorni lavorativi. Si tratta senza dubbio di dati allarmanti che non possono essere ignorati. Si rende necessario, dunque, eliminare inutili vincoli e divieti all'attività d'impresa e rendere più agevole per l'imprenditore il passaggio dalla semplice idea alla nascita dell'attività stessa. Ed è proprio questo l'obiettivo del provvedimento in esame. Per aprire un'attività imprenditoriale, artigianale e commerciale, sarà necessario, d'ora in poi, attendere solo pochi giorni dalla presentazione della domanda di autocertificazione, dopodiché, in assenza di divieti, sarà possibile avviare l'attività. L'idea è buona ed è necessario sostenerla. Non si tratta di una svolta epocale, ma di un piccolo passo avanti nel complesso percorso della sburocratizzazione e della semplificazione amministrativa. Sappiamo bene che il nostro Paese a livello di semplificazione ha sempre incontrato alcune difficoltà, ma questa può essere un'occasione per invertire l'ordine di priorità del complesso rapporto pubblico-privato, facendo in modo che la pubblica amministrazione diventi un alleato dell'attività privata e favorisca la voglia di fare del singolo. Il disegno di legge in esame, oltre all'intento semplificatorio, nasconde in verità un approccio innovativo, in quanto disciplina un'inversione totale del rapporto autorizzazione-controllo: si passa, infatti, da un controllo *ex ante* ad un controllo *ex post.* Se finora l'impresa prima di ricevere l'autorizzazione ad iniziare la propria attività doveva aspettare che venissero effettuati tutti i controlli del caso, con chiare ricadute in termini di tempo e denaro, ora, grazie al nuovo meccanismo introdotto, un imprenditore, attraverso l'autocertificazione e la denuncia di inizio attività, potrà avviare immediatamente la sua impresa che sarà sottoposta solo successivamente ad accurati e severi controlli. Si tratta un approccio nuovo rispetto alla disciplina del vecchio sportello unico che doveva semplificare le procedure, ma che rimaneva, di fatto, nell'alveo delle autorizzazioni preventive. In questo modo sarà possibile evitare tempi morti ed inutili lungaggini. È necessario, inoltre, scongiurare il pericolo che anche questo ennesimo tentativo di sburocratizzazione e semplificazione dell'attività d'impresa resti lettera morta e per questo è auspicabile che le buone intenzioni del disegno di legge in esame si traducano in pratica, fornendo i Comuni italiani delle risorse sia umane che materiali necessarie per dare piena applicazione all'impresa facile. Senza le adeguate risorse finanziarie è difficile, infatti, che i Comuni possano essere in grado di svolgere i compiti che questo disegno di legge loro assegna.

*relatore*. Vorrei osservare che il disegno di legge rappresenta un passo in avanti nella direzione dello snellimento burocratico di cui il nostro Paese ha necessità, soprattutto in relazione all'attività di impresa ancora oggi troppo gravata da costi e da inutili adempimenti amministrativi. La *vexata quaestio* dell'eccessiva burocratizzazione costituisce ancora oggi una grave pecca per la competitività delle imprese italiane e la lotta alla burocrazia rappresenta una questione centrale per rilanciare l'economia del nostro Paese. Di certo questa iniziativa servirà a migliorare la competitività dell'impresa e potrà avere ricadute positive anche in termini di crescita, rendendo il nostro Paese più appetibile anche ad investitori ed imprenditori stranieri. Vorrei ringraziare, infine, i membri della Commissione che hanno condiviso con me le ragioni dello sportello unico. Grazie allo spirito collaborativo che ha caratterizzato i nostri lavori, abbiamo potuto licenziare l'attuale testo, perfezionandolo rispetto alla versione consegnataci dalla Camera di deputati. Ringrazio, inoltre, i funzionari della Commissione per l'ausilio che ci hanno fornito e auspico che il passaggio in Assemblea sia un passaggio costruttivo, un primo ma importante passo verso lo sviluppo dell'impresa italiana.

Il relatore, senatore Pollastri, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

l'Aula è chiamata a pronunciarsi sul disegno di legge n. 1663 concernente la ratifica e l'esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001. L'accordo in esame si colloca nel quadro del rafforzamento delle relazioni tra l'Italia e Cuba ed è volto a regolare nel dettaglio l'esercizio delle funzioni consolari in base alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, in vigore tra i due Stati, posto che negli ultimi anni si è registrato un sensibile incremento degli operatori economici italiani nell'isola, nonché un notevole movimento turistico italiano, oltre che un apprezzabile aumento dei matrimoni misti. In questo quadro si è affermata l'esigenza di provvedere a idonei strumenti di protezione delle persone fìsiche e giuridiche. Giova ricordare che nella scorsa legislatura, pur essendo stato approvato dal Senato il relativo disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, l'esame presso l'altro ramo del Parlamento non è giunto a compimento in ragione delle critiche avanzate dalla comunità internazionale nei confronti del regime castrista nel 2003. Alla luce, tuttavia, del mutato quadro di riferimento attuale si è posta l'esigenza di ripresentare il disegno di legge in esame, che è stato già approvato dalla Camera dei deputati il 21 giugno scorso. Nel merito, la Convenzione presenta una prima parte che si occupa degli aspetti istituzionali della disciplina, regolando lo *status* degli organi consolari, in conformità con i princìpi generali di cui alla citata Convenzione di Vienna. In particolare, si segnala il Capitolo I che in via preliminare precisa il significato della terminologia tecnica impiegata nell'Accordo, mentre il successivo Capitolo II si riferisce alle modalità di istituzione degli Uffici consolari e al procedimento di nomina dei funzionari consolari e degli altri membri del personale Il Capitolo III, infine, regola il regime applicabile in tema di immunità, privilegi e inviolabilità nei confronti di funzionari consolari, nonché di inviolabilità dei locali e degli archivi consolari, prevedendo altresì le condizioni per le esenzioni fiscali e doganali. Si segnala, inoltre, il Capitolo IV che precisa la tipologia delle funzioni riconosciute ai consoli disciplinandone il relativo esercizio. Tra di esse, figurano: la registrazione dei cittadini, il rilascio dei passaporti e dei visti, la notifica di atti giudiziari, la cooperazione in materia di cittadinanza, la legalizzazione di documenti, il rilascio di documenti consolari e l'espletamento di funzioni elettorali, la formazione di atti notarili, gli atti dello stato civile, la protezione dei minori e la competenza nel settore marittimo, la cui disciplina è applicabile - in quanto compatibile anche con riferimento agli aeromobili. In questo quadro, particolare importanza rivestono le norme relative alla libertà di comunicazione tra cittadini e funzionari consolari del proprio Stato, nonché quelle che sanciscono il diritto del console di tutelare i propri connazionali detenuti o comunque privati della libertà. Merita poi segnalare l'articolo 60, che contiene una norma di autorizzazione preventiva concernente l'esercizio di ogni altra funzione consolare attribuita dallo Stato di invio a condizione che tali funzioni non siano in conflitto con la legislazione dello Stato di residenza e che non abbiano ricevuto opposizione da parte delle autorità dello Stato. Di particolare rilievo risulta infine la norma di cui all'articolo 62, che prevede la competenza degli uffici consolari italiani per quanto riguarda l'esercizio di funzioni consolari anche in favore di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che non dispongano di rappresentanze sul territorio. Al Capitolo V, inoltre, si stabilisce che le funzioni consolari possono essere attribuite anche a consoli onorari. Infine, si segnala l'articolo 76, che prevede l'istituzione di una commissione mista, formata da funzionari di entrambe le parti e deputata a vigilare sulla corretta esecuzione delle disposizioni contenute contenute nella convenzione in esame, mentre ai sensi dell'articolo 77 si stabilisce che le eventuali controversie relative all'applicazione ovvero all'interpretazione delle clausole della Convenzione sono risolte per via diplomatica. Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli, rispettivamente concernenti l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria

morì in questo attentato e l'esecutore materiale, Raul Ernesto Cruz, salvadoregno, indicò come mandante dell'attentato tale Luis Posada Carilles, il quale si attribuì,

«La morte del turista italiano è stata solo un incidente imprevisto che non mi turba affatto i sonni. Anzi io dormo come un bambino: l'italiano si trovava nel posto sbagliato nel momento sbagliato». Tale Luis Posada è responsabile di ulteriori attentati, tra cui uno contro un aereo cubano. Egli è stato arrestato e condannato a Panama per avere tentato un attentato contro il Presidente di Cuba Fidel Castro. Nel 2005 Luis Posada Carriles è riapparso negli Stati Uniti, dove è stato fermato per violazione delle leggi sull'immigrazione. L'8 maggio 2007 un giudice statunitense ha dichiarato la liberazione definitiva del terrorista Luis Posada Carriles, non considerando le imputazioni che il Governo degli Stati Uniti aveva presentato contro di lui per frode e per falso nelle dichiarazioni rese al servizio immigrazione doganale del Paese. L'avvocato di Carriles, Eduardo Sota, ha presentato domanda di asilo politico negli Stati Uniti con l'argomentazione

legislazione USA, che afferma che è proibito liberare un sospettato se la sua liberazione minaccia la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, della comunità o di qualunque altra persona, la risoluzione delle Nazioni Unite, approvata dopo l'11 settembre del 2001, precisa che tutti i terroristi devono essere presentati davanti alla giustizia. La morte di questo cittadino italiano attende giustizia da quasi sette anni e il padre di questo cittadino italiano, Giustino Di Celmo, da allora sta combattendo per un diritto che l'onore nazionale dovrebbe tutelare con ogni mezzo.

che l'Italia considera inaccettabile l'eventuale concessione dell'asilo politico al terrorista Luis Posada Carriles e che il trattamento di cui gode un terrorista reo confesso mina gravemente la credibilità dell'impegno degli Stati Uniti nella lotta contro il terrorismo. Si chiede quindi di impegnare il Governo ad adoperarsi con sollecitudine per la richiesta di estradizione in Italia di Posada Carriles nel caso in cui il procedimento penale attualmente in corso presso la procura della Repubblica di Roma portasse a un'incriminazione nei confronti dell'attentato terroristico a L'Avana in cui perse la vita il nostro connazionale Fabio Di Celmo.

che concerne la morte, nel corso di un attentato, del connazionale Fabio Di Celmo. Fu avviato dalla procura della Repubblica di Genova un procedimento penale nel 2000 per il delitto di strage. Questo procedimento fu successivamente archiviato dal giudice per le indagini preliminari con un decreto in data 12 gennaio 2000. Recentemente è stato aperto un nuovo procedimento dalla procura della Repubblica di Roma in ordine al quale il Ministro della giustizia il 15 novembre 2006 ha formulato la richiesta *ex* articolo 8 del codice penale (delitto politico commesso all'estero). Attualmente questo procedimento è pendente ed è contro persone note. Non è stato sino ad ora trasmesso alcun provvedimento restrittivo relativamente al caso appunto della morte di Di Celmo da parte dell'autorità giudiziaria italiana. Questo - come ricordato nel dispositivo - è il presupposto per la formulazione di una richiesta di estradizione. Nel momento in cui l'autorità giudiziaria dovesse emettere un provvedimento restrittivo e il Ministero della giustizia dovesse presentare una richiesta di estradizione, per quanto riguarda il Ministero degli affari esteri si darà immediatamente corso e seguito a tale richiesta.

per annunciare il voto favorevole del mio Gruppo a questa ratifica per l'importanza che assume nella lotta al *doping*, non solo nell'ambito dello sport professionistico, ma anche e soprattutto per la sua drammatica diffusione

Il Ministro della salute è obbligato a rispondere alle interrogazioni. Vorrei sapere quali sono gli strumenti che il Senato mette a disposizione per salvare una vita umana. In questo caso non si parla di coloro che vogliono morire, ma credo che le istituzioni debbono aiutare anche quelli che vogliono vivere. Il caso Steccato è emblematico